la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea. Oggi pomeriggio, alle ore 18, il Ministro dell'interno renderà un'informativa urgente sul caso di Alma Shalabayeva. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno. Nel pomeriggio di giovedì sarà discussa la mozione di solidarietà per l'attività del Ministro per l'integrazione. Venerdì mattina, alle ore 8,30, in luogo del sindacato ispettivo, sarà discussa la mozione di sfiducia individuale presentata nei riguardi del Ministro dell'interno. Per la discussione generale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. La replica del Ministro dell'interno avrà luogo alle ore 10,30. Seguiranno, intorno alle ore 11, le dichiarazioni di voto finale. L'inizio della chiama con appello nominale è previsto per le ore 12,30. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 23 luglio, per 1'esame del decreto-legge in materia di rilancio dell'occupazione e IVA. la giornata dì lunedì 22 sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Restano fermi gli altri argomenti già previsti per questa settimana

2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*** *(Approvato

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato più di un anno e mezzo da quando nel dicembre 2011 il Governo Monti approvava il "decreto salva Italia".

Stiamo discutendo di un provvedimento che sospende per alcuni mesi una tassa che abbiamo considerato ingiusta già nel passato

Dopo aver vessato i cittadini con un'imposta sulle prime abitazioni, sulle pertinenze e sulle imprese, oggi il Governo, con un'inversione ad U, sospende questa tassa sulla prima abitazione fino a settembre; è una sospensione che, però, non risolve in alcun modo il problema e non lo attacca La domanda allora viene fin troppo facile, signor Presidente: dov'è finito quell'impegno, tanto decantato in campagna elettorale, a sostenere le piccole e medie imprese e ad aiutare le aziende? Una indispensabile riorganizzazione deve assolutamente includere anche la questione legata ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D, cioè i fabbricati strumentali alle imprese. lo abbiamo sempre detto, lo continuiamo a dire e lo continueremo a ripetere anche in questi giorni - è una tassa iniqua: è ingiusta e va a sommarsi all'attuale sistema impositivo italiano, il più penalizzante tra quelli dei Paesi dell'OCSE. Signori senatori, ricordatevi questo numero: 68,3 per cento, vale a dire la stima dell'attuale percentuale di imposte e tasse sul reddito che questo Stato chiede alle imprese. Possiamo forse pensare, signor Presidente, che si possa rilanciare il tema del lavoro con una pressione fiscale prossima al 70

a tutti i cittadini la mancanza di attenzione da parte dello Stato nei confronti dei piccoli Comuni, che hanno una grandissima difficoltà a far quadrare i bilanci.

Ben altra cosa era invece l'IMU così come era originariamente pensata, quella prevista nel decreto attuativo delle leggi sul federalismo fiscale:

tassa che per nulla prevedeva una rivalutazione del 60 per cento degli estimi catastali. Signor Presidente, non si è mai visto un periodo così nero: disoccupazione ai massimi da decenni; disoccupazione giovanile oltre il 40 per cento; monte ore della cassa integrazione con picchi altissimi;

Brutte notizie, Presidente! In tutta questa drammatica situazione il Governo blocca per ora il temutissimo aumento dell'IVA e sposta di pochi mesi il pagamento della rata IMU sulla prima casa; e come trova il modo di aggirare e soddisfare il mitico articolo 81 della Costituzione, di cui abbiamo parlato in Commissione e di cui vedremo i danni in fase di approvazione degli emendamenti? Trova la copertura finanziaria con l'aumento degli acconti IRPEF, IRES e probabilmente IRAP:

aziende che ogni giorno combattono la crisi, che cercano di mantenere l'occupazione; aziende che cercano di resistere e lavorare per far sì che tutto il nostro *made in Italy* non venga rastrellato da aziende e imprenditori stranieri.

commissariati, signor Presidente, da questa Europa e da questo asse franco‑tedesco; e pensare che proprio da questi banchi avevamo chiesto al Presidente del Consiglio di rappresentarci in Europa e gli avevamo anche chiesto di battere i pugni sul tavolo per ottenere qualcosa! Abbiamo constatato che il Presidente del Consiglio quel tavolo l'ha appena accarezzato, ha sfiorato e ha raccolto qualche briciola. Sono le briciole quelle che ha portato in Italia! E lei, signor Presidente del Consiglio che non è presente, per quelle briciole ha gridato grande vittoria!

per ragione di competenza personale non intervengo sulla parte fiscale di questo decreto-legge, sulla quale mi limito a proporre un'osservazione elementare: per rimettere in moto un'economia soffocata dal debito e dalla pressione fiscale logica vorrebbe che si destinassero le risorse pubbliche disponibili prioritariamente alla riduzione delle imposte su chi produce (IRPEF e IRAP, lavoro e impresa), in secondo luogo su chi consuma (IVA) e solo in terzo luogo su chi possiede (IMU). L'auspicio di Scelta Civica e il mio è che a queste priorità, sia pure con i compromessi che le promesse elettorali di un partito della maggioranza impongono, si ispiri l'azione del Governo nelle prossime settimane e mesi. Quanto alla parte del decreto dedicata al lavoro, il suo contenuto più rilevante è costituito dal rifinanziamento della cosiddetta cassa integrazione in deroga, essendo altre misure sul mercato del lavoro rinviate al decreto legge n. 76, che abbiamo iniziato a discutere in Commissione oggi. Sulla cassa integrazione in deroga abbiamo sentito questa mattina il relatore Maurizio Sacconi dire che essa ha la funzione di garantire la continuità del legame tra il lavoratore e l'azienda nelle situazioni di crisi temporanea nelle quali il lavoro deve essere sospeso; ripeto: garantire la continuità del legame tra il lavoratore e l'azienda.

Ci terrei che il Sottosegretario per il lavoro mi ascoltasse, perché sto parlando di cose rilevanti per l'economia e per il benessere del Paese... se davvero la cassa integrazione venisse utilizzata, almeno nella maggioranza dei casi per questo scopo, cioè per tenere legato il lavoratore alla sua azienda d'origine, essa svolgerebbe soltanto una funzione utile, perché eviterebbe lo *shock* passeggero che potrebbe altrimenti distruggere capitale umano e destrutturare le strutture produttive. Il fatto è che nel nostro Paese, nonostante le norme legislative che imporrebbero di usare la cassa integrazione soltanto per tale finalità, questo strumento viene attivato sistematicamente anche in situazioni nelle quali è certo ed evidente che i lavoratori interessati non riprenderanno mai a lavorare nelle imprese da cui formalmente ancora dipendono. Quando questo accade, quando cioè la cassa integrazione viene utilizzata per differire il problema fingendo che il rapporto di lavoro prosegua, ovvero nascondendo una situazione di sostanziale disoccupazione, non si fa soltanto un cattivo uso di questo strumento, ma si produce anche un danno grave al lavoratore interessato: lo si tiene infatti legato all'azienda di origine, inducendolo a non attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione, causando in questo modo un allungamento del suo periodo di inattività, di inattività, che a sua volta produce una progressiva riduzione della collocabilità effettiva del lavoratore stesso. Ora, la possibilità introdotta cinque anni fa di erogare la cassa integrazione anche in deroga, cioè in assenza dei requisiti normalmente applicabili per legge, ha sostanzialmente favorito un'ulteriore diffusione del cattivo uso di questo ammortizzatore sociale: esso viene usato oggi in situazioni in cui avrebbe dovuto essere invece attivato il trattamento di mobilità o di disoccupazione. Lo stesso relatore Sacconi questa mattina ci ha detto che in molti casi l'integrazione salariale in deroga è stata erogata a persone che erano già sospese dal lavoro da più di cinque In realtà, l'INPS ci ha recentemente fornito una tabella dalla quale risulta che la cassa in deroga è stata diffusamente erogata anche in situazioni in cui le prestazioni di lavoro erano cessate da oltre sei, sette, otto, nove e addirittura dieci anni e oltre; tutte situazioni, queste, in cui nessuno può ragionevolmente pensare che esista la pur minima possibilità di una ripresa del lavoro nella stessa azienda alla quale il lavoratore viene mantenuto fittiziamente legato per periodi così lunghi. La cassa integrazione in deroga poteva considerarsi un provvedimento eccezionale, e come tale appropriato, all'indomani del fallimento di Lehman Brothers, cioè nell'immediatezza della gravissima emergenza dello scoppio della grande crisi; ma a cinque anni di distanza non può più essere questo il modo in cui si affronta il problema della disoccupazione. La cosiddetta legge Fornero del luglio 2012 indica il modo giusto in cui il problema deve essere affrontato, quello innanzitutto di chiamare le cose con il loro nome: trattare le situazioni di disoccupazione con gli strumenti appropriati. La legge Fornero, oltre a ricondurre la cassa integrazione alla sua funzione essenziale, ha istituito un trattamento di disoccupazione universale di livello europeo, l'assicurazione sociale per l'impiego, che eroga il 75 per cento dell'ultima retribuzione in combinazione con gli interventi necessari per il reperimento della nuova occupazione e sotto condizione della disponibilità effettiva del lavoratore interessato. Le risorse di cui disponiamo dovrebbero essere destinate, semmai, ad allargare il possibile campo d'azione di questo strumento, non della cassa integrazione usata come la stiamo usando, se vogliamo davvero evitare che i nostri lavoratori coinvolti in crisi occupazionali siano destinati a restare per sette, otto, dieci anni congelati nel *freezer* di un trattamento che non ricolloca e non può per sua struttura ricollocare nessuno. Nel nostro emendamento 4.20 al decreto-legge in esame proponiamo che almeno un terzo delle risorse disponibili sia destinato a questo uso, visto che certamente non meno di un terzo dei casi oggi coperti dalla cassa in deroga, anzi presumibilmente molti molti di più, corrisponde a casi di effettiva disoccupazione. Non comprendiamo sinceramente il motivo per cui la Commissione bilancio ha ritenuto di bocciare questo emendamento, che ovviamente non comporta alcun onere aggiuntivo per l'erario. Se questo emendamento deve esser ritirato per esigenze di sollecito varo della legge di conversione, diciamolo e lo ritireremo disciplinatamente per questo motivo, non per un motivo fasullo quale quello di una pretesa incompatibilità con esigenze di bilancio. Chiediamo però che il Governo si impegni a muovere al più presto nella direzione che quell'emendamento e il buon senso indicano, per voltare pagina rispetto a un modo profondamente sbagliato di affrontare le crisi occupazionali, che ha già fatto troppi danni al nostro Paese.

oggi vi parlerò della storia del Grande incendio e della pistola ad acqua usata per spegnerlo, insieme a Nerone, noto per la sua dimestichezza con il fuoco.

per cento su base annua (quindi, più 480.000). Il tasso di disoccupazione si attesta al 12,2 per cento, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a aprile e di 1,8 punti nei dodici mesi (*record* assoluto dal 1977). La cassa integrazione, lo scorso anno, ha sfondato nuovamente - dopo il picco del 2010 - il tetto del miliardo di ore. Calano i consumi, molte famiglie non riescono più a far fronte ai costi delle cure del medico e degli esami, non ce la fanno a pagare le bollette o il riscaldamento di casa. Cresce quindi la povertà, come testimonia l'aumento di persone che si rivolgono alla Caritas, mentre il rischio di esclusione sociale riguarda ormai un quarto della popolazione. Oggi un terzo dei giovani non ha lavoro, e sono in atto oltre 160 crisi industriali. Il potere d'acquisto è tornato ai valori di dieci anni fa, e oltre cinquanta Comuni di media grandezza si trovano sull'orlo del dissesto finanziario. Intanto, la variazione del PIL (diminuito nel 2012 del 2,4 per cento), secondo le previsioni manterrà il segno negativo anche nel 2013. Tra il 2012 e i primi tre mesi del 2013, 121 persone si sono tolte la vita per cause direttamente legate al peggioramento delle loro condizioni economiche. Questo è il Grande incendio che divampa nel nostro Paese, ovviamente con l'aiuto di Nerone. Sono dati conosciuti, ma che è giusto ricordare mentre discutiamo il disegno di legge n. 843: una delle pistole ad acqua che dovrebbero, secondo il Governo, spegnere questo incendio. Le disposizioni previste nel disegno di legge n. 843, di diversa tipologia e natura, danno la sensazione della mancanza di un progetto unitario e di una visione di lungo periodo: si parla di emergenza occupazionale, si parla di ammortizzatori sociali in deroga, si parla di TARSU, di eliminazioni degli stipendi dei parlamentari membri del Governo; tutto mescolato in un unico disegno di legge, dove non si ravvisano misure decisive, soluzioni tali da dare concretezza alla speranza di un cambiamento. Si rinvia il pagamento dell'IMU, la madre di tutte le guerre, la sfida massima che, a quanto pare, questo ambizioso Governo si è posto innanzi. Ben venga la sospensione, soprattutto in previsione di una riformulazione più equa e attenta della tassa. Del resto, le famiglie in condizioni di disagio abitativo sono sempre più numerose:

per finire con l'8,9 per cento che ha difficoltà a pagare le bollette. Ma l'incendio divampa ancor di più tra coloro che la casa non ce l'hanno, o l'hanno perduta; in forte aumento è infatti il numero delle persone che subiscono uno sfratto. Dei 290.000 sfratti emessi negli ultimi cinque anni, ben 240.000 sono per morosità, con la previsione di un incremento di 150.000 nel prossimo triennio; per il 26 per cento sono famiglie numerose, migranti e a basso reddito, e per il 38 per

È proprio la piaga della precarietà a mostrare in tutta la sua gravità il limite delle politiche sociali in Italia. Si finanzia la cassa integrazione in deroga: bene, un provvedimento necessario ed urgente; tuttavia, le questioni vanno affrontate al fine di porre rimedi di carattere strutturale e questo decreto di soluzioni vere non ne trova. In numero assoluto, i precari italiani sono 3.315.580 unità: lo stipendio è mediamente di 836 euro netti al mese (927 euro mensili per i maschi e 759 per le donne). La domanda di stabilità che viene posta dai cittadini e dalle famiglie italiane è chiara, mentre la risposta del Governo risulta insufficiente e confusa; precari, sottopagati, a rischio sfratto, impossibilitati a comprare casa e a mettere su famiglia, defraudati della pensione, ignorati ancora una volta dalla politica, che non vuole vedere e ammettere la necessità immediata e non più procrastinabile di istituire il reddito minimo garantito, riformulando una volta per tutte il sistema degli ammortizzatori sociali. Non so che cosa ancora stiamo aspettando per poter dare questa risposta. Quanto dovrà ancora divampare questo incendio, prima di ammettere che queste pistole ad acqua non sono sufficienti e che Nerone non deve giocare più con il fuoco? Direte che mancano i soldi: non è vero. Siamo capaci di sottrarre soldi alle vittime dei reati di tipo mafioso, ma non di aggredire seriamente gli sprechi della pubblica amministrazione, i costi della politica, la corruzione, l'evasione, recuperando risorse che potrebbero essere reimmesse sul mercato in maniera equa e oculata. Vi ricordo che la spesa complessiva per il finanziamento del *revenu de solidarité active* (RSA) in Francia è una cifra molto simile a quella che l'erario italiano spende per i suoi ammortizzatori sociali. Significa che abbiamo speso per un sistema di *welfare* che tutela solo un lavoratore su due la stessa cifra che in Francia ha garantito a tutti un programma di protezione universalistico e più equo. PRESIDENTE. Senatrice Bencini, la invito a concludere: il tempo sta per scadere. BENCINI *(M5S)*. Bene, allora concludo; concludo con le ultime parole, Vogliamo che ogni lavoratore sia retribuito in modo da garantire un futuro dignitoso a sé e alla propria famiglia. Vogliamo meno ore di lavoro, più persone che lavorano, più qualità di vita, non vogliamo vivere per lavorare ma lavorare per vivere semplicemente e serenamente. È necessario che si formulino quanto prima soluzioni vere e potenti che ridiano fiducia al mondo del lavoro, agli investitori esteri, ai lavoratori e che non siano i soliti palliativi. È necessario che i cittadini ritrovino fiducia nelle istituzioni. Noi crediamo che per essere veramente risolutivi si debbano attuare i principi fondamentali sanciti dagli articoli della nostra Costituzione, unitamente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. europea. È tempo di mollare, quindi, le pistole ad acqua e impugnare l'idrante per affrontare quest'incendio. E visto che...

Grazie. Signor Presidente, colleghi senatori, il mio breve intervento vuole esprimere un compiacimento di fondo sui contenuti del decreto-legge quale segnale di risposta del Governo al popolo italiano su temi sensibili quali la tassazione sulla casa e il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, oltre che sul fronte del contenimento dei costi della politica, più volte richiamato in quest'Aula, concretizzato nell'articolo 3 con riduzione del trattamento economico per gli incarichi di Governo. Voglio rivolgere un invito al Governo affinché si arrivi nei tempi previsti alle decisioni definitive e importanti sulla eliminazione dell'IMU sulla prima casa per le abitazioni principali ad esclusione di quelle di lusso, e non per argomentazioni di natura politica ma solo per alleviare le numerose famiglie italiane dei tanti sacrifici che hanno sopportato per costruire o acquistare la prima casa. La prima casa è il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di costruire la sicurezza del proprio futuro. L'IMU ha indotto preoccupazione nelle famiglie italiane, ansia, timore del futuro; ha fatto precipitare il valore degli immobili ed ha abbattuto gli investimenti nel settore immobiliare; ha dimezzato i mutui erogati alle famiglie nell'ultimo anno; ha ridotto di un quarto in un solo anno le compravendite di abitazioni. Ne è conseguito un crollo per le costruzioni residenziali che ha comportato analoga crisi per altri importanti settori, come quelli dei mobili, degli arredi e delle ceramiche. Si sono così trovati senza lavoro artigiani, fabbri, elettricisti e falegnami, le piccole e medie imprese italiane. Pur consapevole degli sforzi governativi per trovare copertura finanziaria al provvedimento, giova ricordare che aggredire una spesa pubblica sovradimensionata rispetto alla qualità dei servizi offerti può consentire il reperimento di importanti risorse per garantire l'abolizione dell'IMU nell'ambito della complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare. Riforma che potrebbe prevedere per gli immobili sottoposti al pagamento dell'IMU, ad esclusione delle abitazione principali, l'applicazione di costi proporzionali alla migliore classe energetica dell'immobile, per cui chi consuma ed inquina meno avrà minori costi di tassazione. Sarebbe auspicabile anche prevedere misure a sostegno dell'invenduto delle imprese che operano nel comparto dell'edilizia, anche al fine di sostenere un settore vitale per la nostra economia ed evitare che si scarichino i costi sul consumatore finale. In relazione al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, che si aggiunge alla legge n. 92 del 2012, si pongono ulteriori ed oggettivi quesiti sulle possibili modifiche alle disposizioni vigenti e sulla possibilità che si aggravi ulteriormente la situazione occupazionale del Paese, senza che si trovi soluzione alle numerose crisi industriali e lavorative di cui soffrono ampie parti del nostro territorio. È a tutti evidente, infatti, la gravissima situazione di allarme che si sta generando in Italia

Il dato che viene in considerazione attiene alle ingenti somme investite e ripartite tra investimenti comunitari, nazionali e regionali, senza con ciò addivenire ad una ripresa dell'economia e dell'occupazione reale e duratura in favore delle imprese e a salvaguardia del tessuto occupazionale. Né può essere una soluzione quella di spostare sulle imprese la necessità di arrivare al pareggio del bilancio previdenziale elevando l'età della pensione. È invece auspicabile l'avvio di un confronto serrato per affrontare e risolvere il problema del lavoro, ormai drammatica emergenza sociale. Lo sforzo del Governo, dunque, deve essere quello di non trovarsi impreparati di fronte a future misure di contrasto al disagio occupazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e ancora di più dei lavoratori di questo Paese. *(Applausi

la fase di crisi economica in atto, soprattutto la sua persistenza, ci chiama a compiere ogni sforzo per individuare le politiche più opportune per alleviare le difficoltà che le nostre famiglie ed imprese stanno attraversando. Il provvedimento in esame rappresenta un atto con il quale si introducono prime misure volte a fronteggiare questa delicata situazione, al fine di incrementare, da un lato, il reddito disponibile e, dall'altro, i livelli occupazionali soprattutto giovanili. Prima di passare all'esame dettagliato delle singole disposizioni è giusto ricordare l'insegnamento che, sul versante delle *policy*, ci giunge dal più importante economista del secolo passato, John Maynard Keynes. Solo il sostegno alla domanda di beni e servizi, quella comunemente detta domanda aggregata, può consentire alle economie di mercato di uscire da un periodo di profonda e persistente recessione. le misure adottate con il testo che ci accingiamo a licenziare sono volte a sostenere le decisioni di consumo delle nostre famiglie e quindi a stimolare la domanda aggregata. Tuttavia, nel futuro, quando a breve dovremo affrontare un provvedimento di carattere più complessivo, occorre tener presente che, oltre a questo aspetto che oggi stiamo affrontando, ci sono altri elementi su cui dobbiamo concentrare la nostra azione. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito alle Commissioni finanze e tesoro delle Camere i dati relativi alle varie tipologie di unità immobiliari coinvolte nel pagamento dell'IMU e dai dati emerge un'indicazione che dobbiamo tener presente. Nel 2012 da imprese e negozi è arrivato oltre il 40 per cento del gettito IMU complessivo, pari ad oltre 10 miliardi di euro. Nello specifico, la categoria catastale «D», che comprende capannoni, alberghi, case di cura e così via, ha prodotto ben oltre 6 miliardi di euro l'anno, dai negozi arriva

della TARSUTIA e della TARES che le imprese sono chiamate a sostenere in virtù dell'irrisolto problema dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani che nel corso del tempo - e ancor di più in futuro - ha trasformato le imprese in veri e propri bancomat per le casse pubbliche.

senza possibilità di successo la concorrenza dei Paesi emergenti sul lato dei costi del lavoro e dall'altro dei Paesi avanzati con sistemi fiscali più efficienti. La difficoltà a contrarre il costo del lavoro deve spingerci ad adottare tutti quei provvedimenti

il tutto in attesa della riforma (di cui ho parlato poc'anzi) che dovrà affrontare nodi più importanti. Sarà con tale riforma che dovremo rivedere la disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare al fine di renderla meno gravosa per i contribuenti; dovrà rivedere l'attuale disciplina dell'IMU e si dovrà considerare tutto il tema della complessa tassazione e quindi la previsione della deducibilità dell'imposta relativa agli immobili utilizzati per attività produttive dai redditi di impresa. la maggioranza ha tuttavia dimostrato un'attenzione particolare nei confronti delle famiglie italiane fortemente sensibili al tema della tassazione immobiliare in virtù dell'alta quota di nuclei familiari proprietari di un'abitazione. L'attuale crisi economica ha accentuato tale sensibilità, in quanto un numero sempre maggiore di contribuenti incontra delle difficoltà nel pagamento dell'imposta. Ragioni di equità hanno giustificato l'esclusione dalla sospensione di alcune particolari categorie che abbiamo indicato. Nel loro insieme le abitazioni che beneficiano del provvedimento in esame sono quasi 20 milioni e le pertinenze L'estensione del beneficio anche ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali rappresenta un importante aiuto alle imprese agricole, che vedono ridursi il carico fiscale in un momento estremamente delicato per le loro attività. attività. L'esenzione totale dall'imposta con riferimento al patrimonio immobiliare abitativo degli ex IACP rappresenta, dal punto di vista del livello di manutenzione e conservazione del patrimonio, nonché sulle possibilità di sviluppo ed incremento dello stesso, un elemento notevolmente positivo. Sul fronte delle amministrazioni comunali il testo introduce una salvaguardia relativamente alle coperture da garantire ai fini della sospensione dell'IMU. I Comuni sono stati messi in salvaguardia per la rata di giugno in una logica che rispetta le aliquote deliberate dai vari Comuni. In particolare, al comma 2 dell'articolo 1 si modificano le norme sul ricorso all'anticipazione di tesoreria, consentendo ai Comuni di ottenere ulteriori anticipazioni in misura corrispondente al mancato gettito, calcolato sulla base dei dati relativi agli introiti effettivamente incassati nel 2012. Inoltre, al fine di salvaguardare le amministrazioni comunali dagli oneri finanziari derivanti dal ricorso alle suddette anticipazioni di tesoreria, stimati in oltre 18 milioni di euro per l'anno 2013, si è stabilito che gli interessi saranno sostenuti dallo Stato attraverso una serie di misure. misure. Con lo scopo di salvaguardare i conti pubblici e la stabilità delle finanze statali, l'articolo 2 ha introdotto una norma secondo la quale la riforma della tassazione immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013

destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, cioè alla normativa di secondo grado a cui è stata demandata la soluzione di una serie di definizioni e nozioni al fine di rendere efficaci i provvedimenti relativi all'esenzione e alle questioni che attengono soprattutto agli immobili di uso sia commerciale che non. Con questo ordine del giorno si impegna il Governo ad intervenire

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e cari colleghi, farò brevi considerazioni conclusive di questo dibattito perché, come ho anticipato, la richiesta che rinnovo all'Aula è di confermare il testo varato dalla Commissione e precedentemente approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, le considerazioni del senatore Ichino meriterebbero attenzione e, probabilmente, anche norme correttive. Tuttavia, deve prevalere la legittima attesa da parte di molte lavoratrici e di molti lavoratori a che si proceda finalmente, dopo una lunga interruzione, all'erogazione di sussidi mi auguro, sulla base di criteri che saranno oggetto del decreto al quale si fa rinvio nel testo di legge, saranno tali da evitare il ripetersi di quei comportamenti patologici che abbiamo segnalato, in quanto gli ammortizzatori sociali in deroga devono essere orientati principalmente alla continuazione di posti di lavoro che ragionevolmente possono essere nel tempo riattivati e, quindi, alla continuità È ben vero che le politiche passive, che consistono appunto nell'erogazione di sussidi, dovrebbero collegarsi con politiche attive, consistenti cioè in servizi di riqualificazione professionale o di accompagnamento ad una diversa opportunità lavorativa. Ma nel corso di questi anni abbiamo vissuto condizioni davvero straordinarie e penso che nel complesso sia stato giusto dedicare la gran parte delle risorse al sostegno al reddito soprattutto quando questo sostegno al reddito ha consentito la continuazione del rapporto di lavoro. Certo, più colpevole è stata l'assenza di politiche attive quando le Regioni hanno deciso di utilizzare, con le modalità anche smodate che ho segnalato nella mia relazione, lo strumento della mobilità in deroga, che presuppone

la rinnovata intesa con le Regioni che il Governo dovrà redigere quel decreto contenente i criteri di impiego delle risorse, in quella sede anche verificare il collegamento tra politiche attive e politiche passive, soprattutto con riferimento all'utilizzo della mobilità in deroga. Nel provvedimento che esamineremo nei prossimi giorni ci porremo obiettivi di rafforzamento nella rete dei servizi al lavoro, quella rete che comprende tanto servizi pubblici quanto servizi privati, quanto, ancora, servizi di carattere privato o sociale proprio per rendere più effettiva l'aspettativa delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno visto risolversi il rapporto di lavoro lavoro a non essere lasciati soli nella ricerca di una nuova occasione lavorativa. Mi auguro quindi che l'Assemblea del Senato voglia respingere gli emendamenti, di parte dei quali peraltro inviteremo il ritiro, nella convinzione

Vorrei soffermarmi su una puntualizzazione politica da cui non si può prescindere rispetto alle osservazioni che sono state evidenziate. un filo rosso che collega gli interventi della senatrice Paglini e dei senatori Santangelo e Orellana, anche se con sfumature diverse, là dove si sosteneva che la sospensione dell'IMU

La risposta alle prime considerazioni è che quello che viene considerato un elemento di debolezza è invece un elemento di forza. Ci troviamo di fronte al fatto che con la sospensione dell'IMU realizza il primo atto di un processo che poi si svolgerà e che è parte di un quadro complessivo. E noi non dobbiamo perdere il quadro complessivo di riferimento se vogliamo capire qual è il senso di questo provvedimento: non la logica dell'intervento *spot*, non quella della melina, ma il primo passo per una ridefinizione complessiva della tassazione sul sistema immobiliare. Questa è l'altra faccia della medaglia del lavoro che è stato sviluppato in 6a Commissione a cui facevo riferimento nella relazione introduttiva e su cui tornerò fra poco.

in Commissione da questo punto di vista sono stati fatti dei passi avanti significativi con il recepimento di alcuni ordini del giorno. Uno, ad esempio, citato nel suo intervento

con un'intesa dal Parlamento e dal Governo, c'è la possibilità di stabilire come andremo a ridefinire una materia ampia e complessa. Focalizzarci soltanto nel suo punto iniziale non ci permette di vedere il quadro d'insieme e lo possiamo considerare sminuente; ma nel momento in cui invece ne percepiamo tutta l'ampiezza, capiamo che la situazione non è assolutamente questa. Il quadro d'insieme deve essere preso in considerazione sotto molti punti di vista. Il senatore Consiglio, di cui apprezzo sempre gli questa IMU è completamente diversa da quella nata inizialmente. Sicuramente ha subito un'evoluzione, innanzitutto con l'anticipazione che ha avuto con il decreto salva Italia. Mi permetto però di chiedere: ma quel tipo di IMU ha ancora senso nel momento in cui ci rimettiamo mano e dovremo riprendere in considerazione tutto il tema del federalismo fiscale,

nella volontà di non affrontare le cose come tanti *spot* e di cercare di determinare in maniera chiara e semplice l'obiettivo del nostro agire legislativo, ho apprezzato la battuta del senatore Orellana quando ha detto che il titolo del decreto-legge sembrava quello di un *film* della Wertmüller. Su questo concordo penso che dobbiamo ispirarci a quella omogeneità di trattazione normativa che renderebbe assolutamente migliore il tipo di leggi che andiamo a fare. Proprio perché siamo consci di tutto ciò

l'approvazione di questo decreto‑legge serve per dare certezza al diritto e diventa quindi un atto prodromico, un presupposto per la presentazione di un disegno di legge complessivo sulla tassazione sugli immobili che dovrà nascere in un rapporto dialettico con il Parlamento, il lavoro che viene svolto sull'indagine conoscitiva sulla tassazione mobiliare, sapendo che questo è uno dei passaggi. Un altro tema importante, infatti, ha a che vedere con ciò che sta capitando alla Camera dei deputati. Con una rapida approvazione della delega fiscale si andrà ad una ridefinizione degli estimi catastali,

che permetterà questa transizione: una volta approvata la delega fiscale, infatti, avremo cinque anni davanti prima che questa vada a regime e siccome gli interventi che dobbiamo fare sono urgenti non possiamo perdere anche questo come punto di vista importante.

grazie per gli interventi e le repliche. Non posso far altro che confermare quanto è stato già autorevolmente suggerito dai due relatori, senatori Marino Mauro Maria e Sacconi, sottolineando ancora una volta il carattere urgente di questo provvedimento che dà una prima risposta ad alcune caratteristiche caratteristiche negative dell'andamento dei nostri conti pubblici e della nostra economia e che, quindi, richiede una rapida approvazione. serve per dare risposta a coloro che soffrono in aree di crisi per chiusura di aziende e per sospensioni.

tra queste misure urgenti, c'è il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e della mobilità. Sapendo che questo rifinanziamento non sarà sufficiente per far fronte alle esigenze che le Regioni manifesteranno nei prossimi mesi per richieste relative ad ammortizzatori sociali in deroga, ci ripromettiamo di intervenire successivamente con ulteriori rifinanziamenti e aiuti. Ma è importante prendere subito questa decisione e dare la possibilità alle Regioni di utilizzare queste risorse aggiuntive. aggiuntive. Siamo a conoscenza dei problemi che sono nati anche in relazione alla concessione degli ammortizzatori sociali. Non sempre queste concessioni sono state improntate a principi di efficienza e talvolta anche di equità, dovendo affrontare situazioni molto eterogenee sul territorio e facendo riferimento anche ad accordi tra sindacati e Regioni nelle singole Regioni, che spesso adottavano anche criteri diversi per la concessione degli ammortizzatori. D'altra parte, nel decreto-legge è espressamente previsto che il Governo segnatamente i Ministri del lavoro e dell'economia emanino un decreto interministeriale per definire i criteri di concessione. Sappiamo che la Camera ha approvato un emendamento sulla base del quale questo decreto interministeriale richiederà il parere previo delle Commissioni rilevanti dei due rami del Parlamento, quindi avrete la possibilità di intervenire anche in questa fase per dare suggerimenti su come indirizzare quei criteri e uniformarli anche sul territorio nazionale.

Ciò è richiesto dalle condizioni economiche generali, ma anche dalle condizioni politiche che riguardano l'equilibrio all'interno dell'attuale maggioranza. In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, non faccio altro che far mie

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - sull'emendamento 1.0.200 parere non ostativo, nel presupposto che la disciplina transitoria ivi prevista sia riferita esclusivamente ai beni demaniali di competenza statale; sui restanti emendamenti parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, - preso atto delle precisazioni del Governo circa l'adozione di un criterio prudenziale rispetto alla quantificazione della copertura di cui all'articolo 1, comma 4, del testo del decreto-legge, in particolare con riferimento alla prefigurazione del costo di accesso alle anticipazioni di tesoreria nell'ipotesi, pur improbabile, che vi accedano tutti i Comuni; preso, altresì, atto che l'utilizzo degli avanzi di amministrazione consentito dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 non pregiudica le ulteriori somme non vincolate ed il cui utilizzo risulta vietato dall'articolo 187, comma 3-*bis* del TUEL (d.lgs. 267/2000); preso infine atto che il Governo ha assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle esigenze delle Prefetture e delle Questure in materia di immigrazione esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: l'utilizzo delle risorse del Fondo di coesione e sviluppo e di quelle relative al Trattato di amicizia italo-libico, di cui all'articolo 4, comma 1, trattandosi di risorse di conto capitale, comporta una dequalificazione della spesa».

esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.36, 1,40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.0.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.0.200 e 4.26. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti».

si era impegnato, con l'introduzione dell'imposta, tra l'altro con tutto il mondo agricolo, a fare una verifica qualora ci fosse stato un extragettito e, quindi, un introito superiore al previsto, per ritornare poi sulla questione. Abbiamo accertato dai dati che ci sono stati forniti che, per l'anno 2012, vi è stato effettivamente un incremento del gettito. Quindi, con l'emendamento 1.32 proponiamo di tenere fede all'impegno assunto

in ragione della complessità tecnica e del numero ingente di adeguamenti, che, per l'iscrizione prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. del 2011, vi sia una proroga fino al 30 settembre 2013 per consentire di regolarizzare tutte le situazioni. Tra l'altro questa regolarizzazione determinerebbe un aumento di gettito.

La soglia della crisi ci impone di utilizzare strumenti efficaci e definitivi per affrontare e risolvere il dato relativo alla pressione fiscale, che grava sui cittadini come una perenne spada di Damocle. Nel settore agricolo, in tema di imposta municipale propria, il precedente Governo ha adottato strumenti - come ricordato dalla collega De Petris - che non hanno fatto altro che aggravare la crisi in un comparto già fortemente penalizzato anche dal continuo consumo e dall'uso indiscriminato di biocidi.

appare sul piano estimativo non percorribile, in ragione del fatto che i fabbricati rurali, in quanto strumentali all'ordinario svolgimento dell'attività agricola, costituiscono una voce di costo del bilancio agricolo da considerare come avente una rendita catastale pari a zero.

Peccato che non esista un concorso a premi per chi rimanda di più! Noi cittadini abbiamo ribadito più e più volte - e lo ripeteremo all'infinito - che non è possibile continuare a penalizzare questo settore, che è considerato di primaria importanza,

hanno ottenuto una variante, ma che non sono stati inseriti in un piano di utilizzazione aziendale. Ad essi viene imposta l'IMU come se si trattasse, non di terreni agricoli, ma di costruzioni che

di terreni che, avendo una peculiarità, devono essere comunque considerati terreni che hanno già avuto uno sviluppo diverso. di difficoltà che si aggiunge ad un'altra difficoltà: non solo i terreni agricoli vengono penalizzati, ma questi che non hanno una loro definizione vengono ulteriormente aggravati, pur non essendo soggetti ad alcuna espansione di carattere urbanistico, perché l'*iter* attuativo non si è completato.

Dobbiamo stabilire un ordine di priorità. Dobbiamo mettere sul tappeto della nostra agenda politica quello che vogliamo fare e quello che non vogliamo fare, e questo mi pare che sia uno dei temi

Presidente, vorrei in modo particolare riferirmi agli emendamenti relativi alle concessioni demaniali e ai bilanci comunali.

1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.36,

ordini del giorno che sono stati valutati, come dicevo, anche con il Governo e che sono sottoscritti anche da senatori di altri Gruppi politici. Sostanzialmente, si tratta da una parte di un ordine del giorno che impegna che impegna il Governo a normare le disposizioni concernenti le entrate comunali in sede di definizione della legge di stabilità e di rendere possibile, ai fini della predisposizione dei bilanci preventivi, il riferimento alle entrate dell'esercizio precedente. Il secondo propone, propone, attraverso un incremento delle entrate a titolo di maggiori oneri a carico dei titolari di concessioni demaniali marittime a uso ricreativo e turistico, di consentire una risposta all'Unione europea idonea a prevenire la procedura d'infrazione per la violazione che l'Italia già non avendo ancora ridefinito il sistema delle concessioni demaniali, come aveva preso l'impegno di fare entro il 17 aprile 2013.

Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi mi è stata consegnata la relazione del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, relativa alla nota vicenda delle due signore kazake, la mamma e la figlia.

le conclusioni dell'inchiesta interna del Capo della Polizia. Sono qui per riferire di una vicenda della quale non ero stato informato, della quale non era stato informato nessun altro collega del Governo, della quale non era stato informato il Presidente del Consiglio. E sono qui per riferire, attraverso la relazione finale dell'inchiesta interna condotta, come e perché questo sia potuto accadere e cosa occorra fare perché ciò non abbia ad accadere mai più: cioè che un Ministro e l'intero Governo non vengano informati di una vicenda così rilevante. Sono qui per questo. Sono qui a rendere chiaro al Parlamento e alla pubblica opinione quello che è accaduto e per cui abbiamo assunto la decisione, al termine della mia relazione, di mettere sul sito del Ministero dell'interno la versione integrale della relazione di cui mi gioverò nel corso di questo mio intervento. Sono qui anche per ribadire in premessa quanto il Governo ha fatto *post factum*, quanto il Governo ha fatto dopo gli episodi per dare assistenza legale, per continuare ad assicurare il massimo impegno nel seguire con attenzione ogni profilo di protezione internazionale e di salvaguardia dei diritti umani connessi alla vicenda, quello che abbiamo fatto dopo il 2 giugno e ciò che continueremo a fare da questa sera in avanti. L'inchiesta amministrativa è il cuore della ricostruzione della vicenda. Le sue risultanze si compongono di due parti: la prima parte consta di una ricostruzione analitica, giorno per giorno e - dove necessario - ora per ora, di quanto si è verificato; la seconda parte - che è quella che, evidenziando le virgolette, è quella che fa la diagnosi esatta di come sia potuto accadere che il Governo non fosse informato della vicenda. Da questo momento, quello che sto per dire è un virgolettato della relazione finale dell'inchiesta del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza. «Le ricerche «Le ricerche del latitante kazako Ablyazov Mukhtar hanno preso l'avvio nel territorio nazionale il 28 maggio su *input* dell'ambasciatore Adrian Yelemessov. Il processo messo in moto da questa informazione si esaurisce in una fase operativa di polizia giudiziaria consistente in due perquisizioni nella villa di Casal Palocco indicata come nascondiglio del latitante, nel sequestro di denaro, materiale elettronico e di un passaporto, nella denuncia per il reato di falso a carico di Shalabayeva Alma, senza che il Mukhtar fosse rintracciato. Dall'operazione di polizia giudiziaria scaturisce poi un procedimento di natura amministrativa relativo all'espulsione della moglie del latitante. L'incarico affidato allo scrivente è quello di accertare la mancata informativa al Governo sull'intera vicenda che, pur essendo pienamente regolare»,

«Tale incarico quindi è volto essenzialmente ad individuare dove si è fermato il flusso informativo ascendente. È evidente che in ordine alla prima parte della vicenda andrà verificato anche se tutti i funzionari di polizia coinvolti fossero a conoscenza che il ricercato kazako fosse anche un dissidente politico nel suo Paese. È altrettanto necessario che, in ordine alla parte amministrativa dell'intera vicenda, vengano verificate le modalità esecutive dell'espulsione che, al di là della loro chiara legittimità, evidenziano caratteri non ordinari. In primo luogo va ribadito che in nessuna fase della vicenda, fino al momento dell'esecuzione dell'espulsione con la partenza della donna con la bambina, i funzionari italiani hanno avuto notizia alcuna sul fatto che Ablyazov, marito della cittadina kazaka espulsa, fosse un dissidente politico fuggito dal Kazakistan e non un pericoloso ricercato in più Paesi per reati comuni. In nessun momento è pervenuta o è stata individuata negli archivi di polizia informazione che rilevasse lo *status* di rifugiato dello stesso Ablyazov. Anzi, la documentazione fornita dall'ambasciatore kazako, diplomatico ufficialmente accreditato presso il Governo italiano, lo segnalava come elemento collegato alla criminalità organizzata ed addirittura al terrorismo internazionale. In secondo luogo va evidenziato che nel corso dell'intera istruttoria e dalla consultazione di tutta la documentazione fornita non risulta che Shalabayeva Alma o i suoi difensori abbiano mai presentato o annunciato domanda di asilo, pur avendone la possibilità, né è risultato che la citata cittadina kazaka abbia mostrato o affermato di possedere un permesso di soggiorno rilasciato da Paesi Schengen, cosa che hanno fatto i difensori solo in sede di ricorso contro il provvedimento. Al riguardo è opportuno evidenziare che quando per la prima volta Shalabayeva Alma viene condotta presso l'ufficio immigrazione, cioè la mattina del 29 maggio, essa era in compagnia del cognato che, all'atto della verifica della sua condizione di straniero in Italia, affermava di essere titolare di un permesso di soggiorno lettone, quindi rilasciato da Paese Schengen. Nella circostanza veniva verificata la fondatezza dell'affermazione e lo straniero veniva rilasciato. Il tutto accadeva alla presenza della Shalabayeva Alma che avrebbe potuto anch'essa rivendicare la titolarità di analogo documento. Per inciso va rilevato che risultano infondate le affermazioni riportate dagli organi di stampa secondo le quali il citato Seraliyeu Bolat sarebbe stato percosso durante l'irruzione, riportando ferite al volto. Infatti il citato Seraliyeu alle ore 19,20 del 30 maggio si è recato presso l'ospedale Aurelia Hospital ove ha riferito che alle ore 23 del 29 maggio aveva subito una aggressione presso la propria abitazione, cioè nella villa di Casal Palocco, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Si precisa che il predetto è stato fotosegnalato alle ore 18 del giorno 29 maggio e non presentava alcuna lesione facciale e che l'intervento presso la villa di Casal Palocco è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29. La ripetizione della perquisizione, invece, è avvenuta il giorno 31. La ricostruzione della vicenda, esposta cronologicamente sopra», cioè nell'indice cronologico che poi pubblicheremo sul «e convalidata nelle sue fasi dalle competenti autorità giudiziarie, fa ritenere che la prima parte di essa abbia seguito correttamente tutti i circuiti informativi sia discendenti che ascendenti, cioè dal Ministero all'organo procedente e viceversa. La seconda parte, invece, si è fermata nella fase ascendente ad un livello che non ha coinvolto le strutture di diretta collaborazione del Ministro a cui competeva informarlo. Dalla ricostruzione dell'intera vicenda e dalle dichiarazioni acquisite dal vice capo della polizia vicario prefetto Alessandro Marangoni, dal vice direttore generale della Pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale prefetto Francesco Cirillo, da quelle del prefetto Alessandro Valeri, capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, da quelle del prefetto Gaetano Chiusolo, direttore centrale anticrimine, e da quelle del questore di Roma, Fulvio Della Rocca, è possibile ricostruire la seguente cronologia. La mattina del giorno 28 maggio l'ambasciatore kazako a Roma Adrian Yelemessov cerca di contattare inutilmente il Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano. Nella stessa giornata il predetto diplomatico si reca presso la Questura di Roma - Squadra mobile, dove fornisce le indicazioni necessarie per la cattura del latitante kazako Ablyazov Mukhtar, sottolineandone la pericolosità. La sera dello stesso 28 maggio l'ambasciatore fornisce le medesime informazioni al Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno ed al prefetto Alessandro Valeri, capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza. Quest'ultimo contatta il dirigente della squadra mobile che conferma di essere già informato e di aver avviato tutte le conseguenti attività. Il prefetto Valeri informa anche il prefetto Cirillo, a cui fa capo l'Interpol e che svolge tutte le attività già prima descritte ed indicate nell'allegato 1». La relazione è piena di allegati. «Lo stesso prefetto Valeri informa il prefetto Gaetano Chiusolo che a sua volta attiva il Servizio centrale operativo della polizia di Stato, che ha come compito quello di coordinare e seguire le attività delle squadre mobili. Della circostanza viene informato anche il vice capo vicario prefetto Marangoni. L'attivazione duplice delle ricerche del latitante da parte dell'ambasciatore kazako avrà esito negativo e dallo stesso prefetto Valeri verrà data comunicazione al Gabinetto del Ministro dell'interno. A quel momento, come peraltro nei giorni successivi, non era sorto neanche il dubbio che il ricercato fosse un oppositore politico del Governo kazako e che potesse essere oggetto di ritorsioni. La vicenda che attiene al trattenimento ed all'allontanamento dal territorio nazionale di Shalabayeva Alma sembra aver assunto una dimensione rilevante per le autorità diplomatiche kazake. le procedure di espulsione di Shalabayeva Alma sono state eseguite, come è corretto che sia, dalle autorità consolari kazake che sono state solerti nel fornire tutte le indicazioni necessarie all'esecuzione del provvedimento di espulsione ed a rilasciare i documenti necessari per l'espatrio sia di Shalabayeva Alma che della sua bambina Ablyazov Alia. Il coinvolgimento delle autorità diplomatiche kazake non si è però limitato a questa fase ma si è anche sostanziato nell'allertare l'ufficio procedente alla massima attenzione per motivi di sicurezza fino a giungere a mettere a disposizione un volo privato dedicato al trasporto delle due cittadine kazake da Roma ad Astana, capitale del Kazakistan. Anche in questa fase, come sottolinea lo stesso dirigente dell'Ufficio immigrazione della questura di Roma nella sua relazione del 3 giugno, non era pervenuta alcuna informazione che segnalasse rapporti di parentela della donna con un "dissidente politico kazako". Il citato funzionario, primo dirigente della Polizia di Stato, dottor Maurizio Improta, ha dichiarato, come si rileva dall'accluso allegato n. 20, di non aver informato alcuno dei suoi superiori del volo diretto per l'allontanamento della donna, non essendogli stato specificato dal consigliere dell'ambasciata kazaka che il volo fosse appositamente stato predisposto per la stessa. Infatti il funzionario testualmente riferisce:», inizio a leggere il virgolettato del funzionario, «"In ordine all'aereo con cui la donna è stata rimpatriata, va precisato che il 30 maggio, quando ho chiesto la certificazione dell'identità kazaka della donna, il diplomatico presente in ufficio, consigliere Khassen, mi chiese come l'avremmo rimpatriata qualora il provvedimento fosse stato convalidato dal giudice. Nella circostanza spiegai che il rimpatrio sarebbe avvenuto dopo la convalida e anche dopo che ci fossero pervenuti i nulla osta da parte delle autorità giudiziarie competenti. che non essendoci volo diretto per il Kazakistan, avremmo utilizzato la tratta Roma Mosca - Mosca Astana. Nella circostanza il consigliere Khassen ebbe a dirmi che probabilmente, entro qualche giorno, ci sarebbe stato un volo diretto da Ciampino. Lo stesso raccomandava massima cautela perché nel cambio di aereo a Mosca ci sarebbe stato il rischio che uomini armati, pagati dal marito latitante, avrebbero potuto tentare la liberazione della donna. D'altra parte gli "*alert*" sulla pericolosità del soggetto rendevano plausibile tale affermazione. Non diedi seguito alla richiesta essendo ancora necessaria la convalida e l'acquisizione dei lasciapassare. Il giorno dopo, quando lo stesso Khassen venne a consegnare i lasciapassare richiesti conseguentemente alla convalida del trattenimento presso il CIE, il consigliere Khassen mi comunicò che il citato volo da lui precedentemente segnalato era in partenza proprio quel pomeriggio intorno alle ore 17. Comunicò che sul volo erano presenti sia lui che il console kazako e che quindi potevamo anche decidere di effettuare l'espulsione senza scorta, anche perché a bordo c'era personale di volo femminile. Sulla base di questa affermazione non emergeva che il volo fosse stato preso appositamente per il rimpatrio. A questo punto, dopo avere acquisito gli ulteriori nulla osta, incaricavo l'assistente Laura Scipioni di portare i lasciapassare a Ponte Galeria, e insieme al personale che parla la lingua russa, di accompagnare la signora a Ciampino. Nella circostanza, stante le precedenti segnalazioni, chiedo alla squadra mobile e alla Digos, nelle persone dei dirigenti, di coadiuvare ai fini della sicurezza con proprio personale, il trasporto all'aeroporto della Shalabayeva. Non mi risulta che la donna abbia rappresentato all'assistente Laura Scipioni, che parla inglese correttamente, la volontà di chiedere asilo. Non mi risulta che abbia rivolto analoga richiesta all'altro personale, compreso quello che parla la lingua russa. In aeroporto la donna e la sua bambina vengono consegnate, precisamente sotto la scaletta del citato aereo, al console kazako e all'altro diplomatico. In effetti, la consegna alle autorità consolari, invece di avvenire alla discesa dell'aereo in Astana è stata effettuata, sempre alle autorità consolari, in partenza da Roma. Non ho comunicato preventivamente ai miei superiori l'uso del volo Roma Astana, non avendo alcuna possibilità di comprendere che fosse stato l'aeromobile noleggiato appositamente per l'occasione. Non mandando il personale in missione per la scorta della donna, non avevo necessità di chiedere ulteriore autorizzazione"».

Centro Africana difficilmente potevano essere accolte se si considera che si tratta di un Paese per il quale l'UNHCR sconsiglia i rimpatri forzati. Si ritiene opportuno a questo punto ricostruire i singoli passaggi del flusso informativo, che non è pervenuto all'attenzione del Ministro dell'interno. In primo luogo va precisato che il canale informativo che fa confluire le notizie necessarie al Ministro dell'interno è di norma il Capo Gabinetto del Ministro o direttamente il Capo della Polizia, oppure i loro sostituti. Gli uffici sui quali si concentra il flusso informativo che fa riferimento al Capo Gabinetto è l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, quello che fa riferimento al Capo della Polizia è la segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza. È evidente che non tutte le informazioni sono portate a conoscenza del Ministro in quanto sono preventivamente selezionate in ordine di importanza e rilevanza. Tale valutazione compete ai vertici dei citati uffici che, sulla base dell'esperienza, della prassi, delle esigenze, delle circostanze contingenti e del contesto generale, classificano le informazioni secondo un ordine di priorità a cui sono collegati comportamenti conseguenti. Per quanto concerne le espulsioni ai sensi della normativa vigente, le stesse, che sono predisposte con provvedimenti dei prefetti, non vengono assolutamente segnalate al Ministro che ne può prendere tutt'al più cognizione periodica sul piano meramente statistico. Nel caso in esame è evidente che nella prassi non esisteva obbligo di informazione al Ministro, sia perché si trattava di un'espulsione ordinaria, sia perché non vi era né evidenza, né consapevolezza che il marito della espulsa fosse un dissidente, sicché nessuna informazione è stata data al Ministro. Va di converso detto che l'attenzione di un altro Paese così evidente e tangibile attraverso l'impegno diretto del proprio ambasciatore e l'utilizzo di un volo non di linea per il rimpatrio delle due cittadine kazake, avrebbe dovuto rappresentare elemento di attenzione tale da far valutare l'opportunità di portare l'evento a conoscenza del Ministro

dai vertici del Dipartimento della Pubblica sicurezza al Gabinetto del Ministro. È mancata in quel momento però l'attenzione ad una verifica puntuale e completa su tutto il rapporto innescato dalle autorità diplomatiche kazake che avendo coinvolto direttamente il Gabinetto del Ministro avrebbero dovuto essere seguite in tutte le fasi del loro rapporto con gli organismi territoriali, a cui è demandata la mera operatività. Non è stata seguita per niente dal Dipartimento della Pubblica sicurezza la fase relativa all'espulsione della moglie del ricercato, a cui gli organi territoriali hanno attribuito un mero valore di ordinarietà burocratica, come la si evince anche dal tipo di coinvolgimento della prefettura di Roma che ha predisposto il provvedimento di espulsione, la cui richiesta è pervenuta ordinariamente via fax e senza sollecitazioni o particolari avvertimenti. Il punto nodale della ricostruzione quindi è comprendere perché si sia fermato il flusso informativo che fino a un certo punto ha coinvolto la segreteria del Dipartimento e il Gabinetto del Ministro e nella fase conclusiva si sarebbe bloccato a livello di uffici territoriali. In effetti il questore di Roma, sentito dallo scrivente nell'ambito della disposta inchiesta amministrativa, afferma di non avere dato direttamente informazione al Dipartimento nelle varie fasi dell'attività svolta dai suoi uffici, perché consapevole che lo stesso Dipartimento fosse direttamente informato dagli stessi uffici della questura. Su questo punto si è soffermata l'attenzione dello scrivente, in quanto anche qui emerge la differente gestione delle due fasi della vicenda: quella delle ricerche del latitante e quella dell'espulsione della moglie. Dagli atti assunti si ha precisa informazione della correttezza del flusso informativo sino a quando si acclara l'esito negativo delle ricerche di Ablyazov. Per quanto riguarda le fasi successive, il prefetto Valeri ha memoria solo delle informazioni relative alla fase di polizia giudiziaria ma non ricorda quando ha appreso dell'espulsione della donna e delle modalità esecutive dell'espulsione stessa. Il dirigente dell'Ufficio immigrazione, che ha mantenuto i rapporti con gli organi investigativi territoriali, Squadra mobile e DIGOS, non ha attivato canali autonomi di informazione né nei confronti del questore né del Dipartimento della pubblica sicurezza, non avendo percepito la straordinarietà delle modalità con cui l'espulsione è stata eseguita. In termini conclusivi emerge che il Dipartimento della pubblica sicurezza non ha seguìto in tutte le sue fasi il processo stimolato dalle autorità diplomatiche kazake che avrebbero voluto investirne direttamente il Ministro ma che erano riuscite a raggiungere solo il suo Capo Gabinetto. Lo stesso Dipartimento della Pubblica sicurezza ha seguito l'evolversi delle iniziative dei diplomatici kazaki solo fino a un certo punto, come se dovesse rispondere al Gabinetto del Ministro solo relativamente all'eventuale cattura del latitante e non dell'insieme dell'operazione. Tanto si rassegna per i provvedimenti che la Signoria Vostra intenderà adottare». Chiuse le virgolette. Per quanto riguarda i provvedimenti che si intendono adottare, dicevo, sono qui per rendere conto di una vicenda della quale non sono stato informato e della quale il Governo non è stato informato. del Governo, nel comunicato del 12 luglio, la regolarità formale del procedimento e la sua base legale sono state accertate e convalidate da quattro distinti provvedimenti di autorità giudiziaria di Roma: procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni il 30 maggio, giudice di pace il 31 maggio, procura della Repubblica presso il tribunale e procura della Repubblica per i minorenni il 31 maggio. A questi provvedimenti si deve aggiungere l'indagine avviata dalla procura di Roma nei confronti della signora Alma Shalabayeva, al cui ambito appartiene il provvedimento di dissequestro del giudice del riesame concernente il denaro e la *memory card* sequestrati alla signora. Tuttavia - è quello che dicevamo, è quello da cui è scaturita l'inchiesta interna e ciò per cui assumo delle decisioni - resta grave la mancata informativa al Governo sull'intera vicenda che, comunque, presentava fin dall'inizio elementi e caratteri non ordinari. ordinari. Noi dobbiamo lavorare perché ciò non accada mai più. Allora, ho chiesto al Capo della Polizia, al Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, una riorganizzazione complessiva del Dipartimento stesso, a cominciare dal vertice del settore immigrazione, cioè della Direzione centrale dell'immigrazione. accettato - e l'ho fatto con profondo rispetto per la sua carriera onorabile di brillante funzionario dello Stato - le dimissioni del mio Capo di Gabinetto ed ho proposto l'avvicendamento del capo della segreteria

della pubblica sicurezza e una riorganizzazione complessiva del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui contenuto non è competenza del Ministro entrare. Tuttavia, ho chiesto al prefetto Pansa di farmi avere quanto prima una sua proposta di riorganizzazione generale. A questo si affianca l'azione inesausta che il Governo porrà in essere nei confronti del Governo del Kazakistan per assicurare che i diritti umani non vengano violati e che, qualora ci siano le condizioni, le cittadine kazake possano essere libere di tornare in Italia. È questa l'azione che sta svolgendo il ministro Bonino e che ha svolto l'intero Governo.

non accada mai più e che mai si possa dire che un Ministro e un intero Governo non siano a conoscenza di quanto accaduto. Tutto questo lo dico nel profondo rispetto, che voglio ribadire a questa

durante le dichiarazioni del ministro Alfano ho visto, ahimè, veterani della fibrillazione rigirarsi sul loro scranno ed anche i tanti neoassunti a questa non illustre professione avere delle difficoltà sul come proiettarsi verso i passaggi dei prossimi giorni (mozioni di sfiducia ed altro). La prima cosa che si può rilevare è il profondo senso delle istituzioni, la compiutezza delle informazioni, la velocità con la quale le stesse sono state fornite e con la quale si è promesso di metterle a disposizione

Nella sua relazione il ministro Alfano ha precisato che il kazako viene aggettivato più volte come «latitante»

i kazaki hanno preso l'iniziativa di denunziarlo alla questura (iniziativa giuridicamente valida) e hanno preso la decisione politica di portare tale denunzia ai livelli più alti della politica, ossia al Ministero dell'interno. notiamo però una manchevolezza, che viene avvertita da chi, meglio di noi, si occupa del settore. Perché l'azione dell'Interpol doveva essere doverosamente coordinata non soltanto dal Dipartimento della pubblica sicurezza,

di questo però non ci può essere una responsabilità, perché non si può parlare in modo virtualmente valido di responsabilità oggettiva. Ottimo è stato il comportamento del Governo, lampante è la sua estraneità, altrettanto lampante è il fatto che non ci si può ricondurre a una

essere molto soddisfatti delle dichiarazioni del ministro Alfano e lo invitiamo a procedere nella sua azione e nella sua attività politica.

Signor Presidente, poche ore fa il capo di Gabinetto del ministro Alfano, Giuseppe Procaccini, si è dimesso. È presumibile, come è stato detto anche in quest'Aula, che nelle prossime ore si aggiungeranno alle sue altre dimissioni altrettanto autorevoli. L'intera linea di comando del Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale sembra essere coinvolta nell'operazione che, come è stato ricordato, negli ultimi giorni del maggio scorso portò a quello che noi chiamiamo sequestro illegale e al rimpatrio di Alma Shalabayeva e di sua figlia. Tutti tranne il vertice della piramide, il Ministro dell'interno. È credibile questo? È possibile cioè che un'operazione di tale importanza e delicatezza sia stata decisa, organizzata e portata a termine senza mettere al corrente il responsabile numero uno del Ministro dell'interno? Anche se si volesse dare a tutti i costi una risposta positiva, nonostante i molti elementi che attestano il contrario, è credibile che un Ministro non si accorga di niente, mentre sotto i suoi occhi viene portata a termine un'operazione di queste dimensioni, e continui a ignorare tutto nelle settimane e nei mesi successivi? In un caso come nell'altro, a nostro avviso, quel Ministro non può restare al suo posto. Quell'operazione, va ricordato, fu portata a termine in tempi fulminei (appena 48 ore) e con grandissimo dispiego di mezzi e uomini (almeno 50 agenti parteciparono all'azione), violando ogni regola, al punto da rispedire le persone rapite - di questo si è trattato, di un rapimento nel loro Paese con un aereo privato noleggiato dal Governo del Kazakistan. È plausibile che tutto questo sia stato fatto tenendo il Ministro all'oscuro? Il 28 maggio l'ambasciatore kazako incontrò al Viminale il Capo di Gabinetto, che lo ricevette al posto del ministro Alfano, cui era stato chiesto in prima battuta il colloquio, come lui stesso ci ha detto. Fu in quella occasione che fu deciso il *blitz* scattato poche ore dopo. Qualcuno davvero può credere che lo stesso Ministro non sia stato informato quando si usano 50 uomini, - lo sottolineo, 50 uomini - per un'operazione di polizia? È normale, Ministro, utilizzare 50 uomini per quella che lei ha definito una normale espulsione? Del resto, di elementi incredibili questa storia, che copre di vergogna il nostro Paese, ne presenta fin troppi, e non riguardano solo il Ministero dell'interno, ma anche il Ministero degli affari esteri, già protagonista, pochi giorni fa, dell'increscioso e a tutt'oggi inspiegato episodio della chiusura dello spazio aereo nazionale, che io stesso ho più volte sollevato in quest'Aula, per il volo del presidente boliviano Evo Morales. Il 30 maggio, subito dopo questa *rendition*, che è persino più grave di quella già intollerabile di cui fu fatto oggetto Abu Omar, la Farnesina dimentica di segnalare all'ufficio immigrazione che Alma Shalabayeva è moglie di un importante dissidente kazako e nella stessa giornata il prefetto di Roma firma il decreto di espulsione a carico della donna, attribuendole precedenti penali in realtà inesistenti. Il 31 maggio l'ambasciata kazaka invia un fax all'ufficio immigrazione della questura di Roma per complimentarsi della brillante e soprattutto celere operazione. Neppure in questo caso, Ministro, secondo le ricostruzioni ufficiali, viene fatto a lei alcun cenno del fax e tanto meno dell'operazione per cui arrivavano tanti e così meritati complimenti. Ci dispiace dirglielo, ma davvero stentiamo a crederlo. Il 5 giugno però, Ministro, lei - che pure dell'intera faccenda dice di non sapere niente - si sente in grado di garantire che tutte le procedure sono state correttamente rispettate. Da quel momento il Ministro, secondo la versione ufficiale dei fatti, torna però a dimenticarsi dell'accaduto e per quasi 40 giorni dimentica di fare luce su un episodio gravissimo che, se davvero si fosse verificato a sua insaputa, egli avrebbe dovuto ritenere ancora più intollerabile, com'è del tutto evidente. Questi sono solo alcuni degli elementi oscuri che gravano su questa vicenda Non vogliamo unirci al coro numeroso dei dietrologi, ma è difficile non sospettare che dietro questa solerzia dell'intero apparato della pubblica sicurezza e a queste clamorose violazioni dei diritti umani e delle stesse leggi dello Stato ci siano non soltanto errori di valutazione, ma la difesa di interessi precisi, legati forse alle fonti energetiche del Kazakistan. Ma non è questa la sede per affrontare questo tema, perché non vogliamo fare dietrologia. Qui si discute semplicemente delle eventuali responsabilità di un Ministro della Repubblica in una vicenda che ha ferito la dignità e l'onorabilità della Repubblica stessa. Diciamo le cose come stanno: tutto porta a concludere che in queste ore il ministro Alfano e con lui l'intero Governo si stiano dando da fare per trovare capri espiatori a cui far pagare le loro responsabilità. Al Parlamento e all'intero Paese viene consegnata una verità tanto rassicurante quanto falsa: nessuna responsabilità politica, solo funzionari scorretti e incapaci, che sono stati tempestivamente individuati, colpiti e rimossi. Peraltro, non è certo la prima volta che un *leader* politico cerca di coprire le proprie responsabilità chiedendo al al Parlamento di avallare una storia incredibile - diciamo così - anche a costo di coprirsi di ridicolo in nome della convenienza e della difesa di una maggioranza. È successo recentemente quando Silvio Berlusconi ha inflitto un colpo micidiale alla credibilità delle istituzioni democratiche chiedendo ai parlamentari della sua maggioranza di avallare la versione fantastica di Ruby nipote di Mubarak. *(Applausi dal Gruppo

Noi speriamo che oggi non ci si presti allo stesso gioco e non si contribuisca ad affossare la credibilità del Parlamento e delle istituzioni solo perché, a differenza di qualche anno fa, è cambiata la collocazione politica. Ma come ho già detto, dal punto di vista delle conclusioni, credere o meno a questa versione per noi cambia davvero poco. Se anche fosse vero che tutto si è svolto sotto gli occhi del Ministro senza che lui si accorgesse di niente,

poche settimane fa, per motivi infinitamente meno gravi, l'allora ministro Josefa Idem scelse la via della dignità e dell'assunzione di responsabilità e lasciò volontariamente il suo Dicastero. Sarebbe davvero inaccettabile se oggi, per un episodio di ben maggiore rilevanza, il ministro Alfano restasse invece al suo posto.

con documenti regolari, vengano espulse e poi rimpatriate con queste modalità ci imbarazza.

C'è un minore che è stato praticamente rapito, deportato - sono parole forti, ma questa è la realtà

La stampa ci riferisce di sollecitazioni ad intervenire esercitate direttamente sulle istituzioni italiane.

come tale è stata valutata poi nel merito da altri esponenti del Governo in carica nonché dal tribunale del riesame in seconda convalida. Risulta peraltro inverosimile la giustificazione addotta dal Ministero degli affari esteri circa l'essere stati indotti in errore a causa del cognome da nubile della signora, dato che la richiesta di verifica sul passaporto è avvenuta soltanto dopo il *blitz* nell'abitazione della donna. Se fosse realmente questa, signor Ministro, l'imbarazzante giustificazione della Farnesina, ci troveremmo di fronte ad una manifestazione di pericoloso dilettantismo. *(Applausi dai Gruppi sarebbe ipotizzabile una condotta in malafede da parte di elementi del personale del Ministero.

Come faceva il Governo Letta a non essere informato su un'operazione così delicata? Questi sono i chiarimenti che dovete dare. quale motivo sono stati calpestati i diritti fondamentali di *status* e di protezione diplomatica della signora e della figlia di sei anni?

Signor Ministro, dalle sue parole cogliamo il profondo rammarico per non essere stato informato di questa grave vicenda e la consapevolezza della profonda serietà di questo delicato passaggio per la vita delle nostre istituzioni, nonché di una inquietudine diffusa nel Paese e in tutti noi per un episodio che fa precipitare nuovamente il nostro Paese nelle notti più buie della storia della Repubblica. È infatti inaccettabile che una delle maggiori democrazie del mondo abbia al suo servizio - si fa per dire una burocrazia nei confronti della quale lei ha usato parole molto severe, che noi apprezziamo, e che si rende protagonista di episodi tanto agghiaccianti. Non le sfuggirà, signor Ministro, che episodi simili compromettono la nostra credibilità sul piano internazionale e ci relegano ai margini delle Nazioni più virtuose in tema di diritti umani e civili, come purtroppo anche analisi internazionali hanno più volte riaffermato. Ma ciò che è più inquietante è la convinzione, che pervade evidentemente larghi settori degli apparati di sicurezza e di difesa, di essere al di là della legge, sottratti alla direzione della politica, quasi impunibili rispetto ad atti e fatti che, se solo fossero oggetto di un'approfondita meditazione, non sarebbero certo commissibili. Scelta Civica per l'Italia, signor Ministro, coglie dalle sue dichiarazioni e dalla relazione che ha ricostruito questa triste ed inquietante vicenda, che approfondiremo, ogni spunto spunto per poter esprimere una più compiuta valutazione, ma giudica positivamente e come dovute le dimissioni già rassegnate, che tuttavia non sono sufficienti rispetto all'estrema gravità dei fatti. evidenzia l'importanza dei provvedimenti che lei ha già annunciato e la necessità di fugare ogni dubbio su possibili subalternità, soprattutto nei confronti di Paesi con i quali abbiamo non secondarie relazioni economiche, ma che sono riprovevoli dal punto di vista dei diritti civili ed umani. Scelta Civica seguirà l'evoluzione che la vicenda probabilmente avrà nei prossimi giorni e venerdì trarrà le proprie conclusioni sulla mozione presentata, invitando comunque lei, signor Ministro, ed il Governo nel suo insieme, a mettere davvero in atto tutte le iniziative già annunciate, di carattere amministrativo,

in questa sede lei è venuto a raccontare una grande menzogna e la pessima trama di un film nero di serie Signor Ministro, la grande menzogna è che nella notte del 29 maggio si stesse cercando un ricercato: non è vero non è vero e non lo diciamo noi. Lo dice una risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2013 - del quale si poneva già l'attenzione sul comportamento del Kazakistan, che era uso perseguitare i familiari degli oppositori politici, e si metteva in guardia il nostro e gli altri Paesi da questi comportamenti,

che il 21 dicembre 2012, a seguito della causa avviata il 20 novembre 2012 dal procuratore generale del Kazakistan, il tribunale distrettuale di Almaty ha messo al bando il partito

cioè il partito del marito della signora Shalabayeva: quello che lei definisce un ricercato, era dunque il capo del principale partito di opposizione del Era un esule politico, signor Ministro, riconosciuto tale dal Governo inglese. La grande menzogna che si menzogna che si viene a dire in quest'Aula, signor Ministro, è che si cercava un ricercato, mentre le intenzioni erano chiare. Quando un Governo noleggia un aereo privato dal costo di 100.000 euro al giorno e lo porta a Ciampino, non aspetta un ricercato, perché come lei sa, signor Ministro (e non può certo venirci a dire qui il contrario), un ricercato con mandato di cattura internazionale, qualora fosse trovato dalle nostre forze di polizia,

L'avrebbe atteso invano. Lo sa perché, signor Ministro? Perché i Paesi europei non estradano nessuno, neanche i peggiori criminali, verso il Kazakistan. Ci sono diverse pronunce verso veri criminali che non sono stati estradati. Lo sa perché, signor Ministro? Perché le convenzioni internazionali, la normativa europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo impediscono di estradare perfino i criminali: non una madre o una bambina di sei anni, ma i criminali non possono essere estradati verso un regime come quello kazako! Lei, signor Ministro, ci viene a raccontare adesso che non sapeva e che non ne era a conoscenza: questa non è una storia credibile. È la trama di un film di serie zeta che nostri funzionari di polizia abbiano tradito il loro compito. Non è così, signor Ministro: essi hanno agito

il dittatore del Kazakistan va a fare le vacanze non nelle ville di quei funzionari di polizia, ma nelle ville dei sodali del signor Berlusconi. Non ci venga a raccontare storie! *(I senatori del Gruppo M5S si Ministro, per le sue responsabilità, con gli uomini in divisa che difendono la libertà in questo Paese e che hanno seguito i suoi ordini, probabilmente senza capire quello che facevano o per compiacere il suo Ministero e chissà chi altri. lei deve compiere un atto di responsabilità che dia uno straccio di dignità a questo Paese, che con il suo operato lei ha buttato nel fango. Il suo Ministero ha infangato il nome dell'Italia, ha messo a rischio una donna e la sua bambina,

in quale Paese pensa di vivere? In quale Paese civile, democratico e occidentale una madre e una bambina possono essere consegnati

signor Ministro,

prima ancora che agli organi di informazione, nel rispetto delle istituzioni parlamentari e accogliendo le sollecitazioni che erano venute dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato e, ritengo, anche dalla Camera, dove dopo questa informativa si recherà.

Comprendo - e non me ne meraviglio, avendone viste tante nella vita - anche l'enfasi dello scontro politico che alcuni vogliono alimentare. Del resto, parliamo del Kazakistan, un Paese certamente controverso, la cui identità politica democratica è tutta da definire,

ciò non vieta alla nomenclatura mondiale di incontrarlo, stringergli la mano e confrontarsi con lui. Che poi il Kazakistan debba guadagnarsi credenziali credenziali di credibilità democratica nel contesto internazionale lo sappiamo bene e non lo scopriamo oggi. Quindi, se il *leader* kazako è certamente personaggio al centro di mille polemiche e discussioni,

dove scrivere gli uni o gli altri, a cominciare anche dalle autorità del Governo kazako, ma vale anche per il personaggio di cui si parla, Ablyazov, e i suoi familiari. familiari. Probabilmente è il capo dell'opposizione, un dissidente, non lo so, ma è anche un personaggio al quale nel Regno Unito, nella democraticissima Gran Bretagna, sono stati sequestrati ingenti beni, per diversi miliardi non so se di dollari, euro o sterline. o sterline. Certamente, però, ingenti risorse sono state sequestrate a questa persona, sono state addirittura messe in vendita, quindi ci sono atti realizzati in molti Paesi nei confronti di questo personaggio, che probabilmente non è Garibaldi. Non sono in grado di trarre conclusioni, non ho strumenti investigativi che mi possano far dire chi sia in realtà Ablyazov. Nel passato, da quel che si è letto nelle cronache, è stato collaboratore di Nazarbayev, esponente che aveva avuto una possibilità di crescere nel mondo imprenditoriale e bancario di quel difficile e controverso Paese. Può darsi che sia un dissidente o uno speculatore. Quello che sappiamo è che l'Interpol ha emesso ordini di cattura avallati da più Paesi, non solo dal suo Paese originario, dove si potrebbe immaginare una ritorsione, una vendetta o un contrasto, se fosse soltanto un dissidente. Potrebbe esserlo (chi lo sa?), ma è ricercato da organi investigativi internazionali. Da questo, infatti, bisogna partire: il dipartimento di pubblica sicurezza, la questura, gli organi che sono stati puntualmente richiamati nella relazione che il Ministro dell'interno ha svolto (e che a sua volta egli ha ottenuto dal capo della Polizia Pansa, citato

Paese che - come ha ricordato il ministro Alfano, vice Presidente del Consiglio, ma già lo sapevamo avendolo letto sulle cronache giornalistiche - quattro distinti provvedimenti dell'autorità giudiziaria

assunti le responsabilità, ma sulla base di un avallo della magistratura di questo Paese, della procura della capitale d'Italia e quindi senza arbitri. Poi, ripeto, che fossero perseguitati o altro è tutto da vedere. Come è stato ricordato anche qui, la signora Shalabayeva non ha chiesto l'asilo diplomatico. Si è parlato della Repubblica centroafricana: ho letto sui giornali, ma non so se sia vero, che la signora nel passato era stata proposta come console del Burundi. Ora, non so se questi erano modi per sfuggire a persecuzioni kazake o per coprire attività più o meno ambigue di questa famiglia. Come ha ricordato il Ministro dell'interno poco fa, in Paesi come la Repubblica centroafricana viene sconsigliato da organismi internazionali di instradare Non sono un investigatore e non sono in grado di sciogliere questi misteri, ma ce ne sono tanti. Probabilmente, alcune circostanze saranno state sottovalutate dagli uffici competenti, è possibile, e siamo qui del resto a discuterne nel Parlamento della Repubblica alla presenza di buona parte del Governo

Alfano è chiarissima e piena, a maggior ragione per l'annuncio di questa riorganizzazione che è stato fatto dal Ministro dell'interno, e anche nell'apprezzamento di funzionari

che nel Regno Unito e in altri Paesi hanno visto protagoniste queste persone, il fatto che, quando il cognato di questa signora ha potuto mostrare credenziali della Lettonia, immediatamente le autorità di polizia ne hanno preso atto e hanno consentito la sua permanenza in Italia,

non solo alcune Repubbliche asiatiche, ma anche Paesi dell'Occidente intervenire con durezza e con determinazione. La ringraziamo, quindi, ministro Alfano, per la ricostruzione che ci ha offerto questa sera. Ne traiamo anche noi, come parlamentari, elementi di riflessione per verificare leggi, rapporti internazionali e organizzazioni diverse che lei stesso ha annunciato. Rifiutiamo, però, ogni tipo di speculazione politica: se qualcuno ha altri intenti, lo dica con chiarezza. Noi vogliamo che il Governo, anche per garantire la sicurezza dell'Italia, prosegua la sua azione; chiediamo che lo faccia nella sua interezza, quindi con il vice presidente del Consiglio e ministro dell'interno Alfano, che ringraziamo per quanto ci ha detto e che potrà contare sul nostro leale, totale, pieno sostegno.

facile, signor Presidente: di queste comunicazioni. Anche noi, come altri hanno fatto, sottolineiamo che investire da subito il Parlamento, prima che incominci l'esame al microscopio della relazione sulla stampa, è una cosa importante e giusta. Prendiamo atto del suo intervento intervento e del dato essenziale contenuto nella relazione, che lei ha riferito, ossia che la catena che si è sviluppata non è giunta ad informare il Ministro. Ci riserviamo un approfondimento doveroso di tutti gli elementi informativi che lei ci ha consegnato, che sono tanti e meriteranno sicuramente uno scrupoloso studio da parte di tutti. L'informativa che ci ha dato descrive una vicenda anomala, grave e inammissibile in un Paese come il nostro. Non mi fermerei ai dati burocratici; guardiamo in faccia la realtà: questo è un atto che ha dato e da un colpo serio all'immagine del Paese, e noi non ne avevamo bisogno in questo momento in cui l'Italia tutta, e il Governo in prima persona, stanno attuando un grande sforzo per ridare credibilità al nostro Paese. Nelle cose che lei ha detto, signor Ministro, sono chiamati in causa temi, questioni e valori di principio rilevanti in ogni democrazia matura. Innanzitutto la tutela dei diritti umani, sempre e comunque e ancor di più quando ci sono di mezzo donne e bambini, e il nostro pensiero non può non andare, appunto, alla situazione della signora Shalabayeva e di sua figlia, che non possono essere considerate mere annotazioni in un rapporto. Vi sono poi l'efficacia e la proporzione delle azioni di polizia, come giustamente è stato ampiamente esaminato, il modo di gestire le informazioni, la catena dei ruoli e delle responsabilità dentro le strutture dello Stato, fondamentali esigenze di trasparenza. Di tutto questo lei ci ha parlato e di tutto questo siamo investiti: sono tutte questioni grandi e delicatissime, che non possono concludersi con esiti incerti o incompleti. Prendiamo atto di tutti gli elementi che già ci sono e sin d'ora chiediamo a lei e a tutto il Governo che si tengano accesi tutti i riflettori sulla vicenda, non si risparmino energie nell'andare fino in fondo e nel seguire tutti gli eventuali sviluppi, perché non è detto che questa vicenda abbia finito di dire cose, verità e magari anche qualche mistero. Gli interrogativi sono tanti, tanti ne ha posti lei, o a tante risposte ad interrogativi ci ha chiamati lei, e a molti di essi la relazione dà risposta, ma tanti altri abbisognano di ulteriori approfondimenti, come afferma la stessa relazione lei ha letto; ci riserveremo anche noi di segnalarli non appena avremo avuto modo di approfondire. Alcune questioni restano per noi bisognose di approfondimento. perché le autorità diplomatiche kazake possono rivolgersi alle nostre strutture di polizia con tanta dimestichezza e diretta relazione? Perché l'attenzione spasmodica sulla famiglia delle stesse autorità non ha destato sospetti e qualche elemento di intelligente e pronta risposta? A che punto è oggi il nostro confronto con le autorità kazake dopo la vicenda che si è verificata? Sono questioni che abbisognano di ulteriori approfondimenti, e chiediamo al Governo di tenere costantemente informato il Parlamento di ogni evoluzione. Un altro aspetto decisivo è in questo caso quello delle responsabilità. Occorreva che vi fossero sanzioni, e lei ce ne ha comunicate alcune, provvedimenti disciplinari esemplari commisurati alla gravità della vicenda. Non è il bisogno di capri espiatori ma la fisiologica necessità di ripristinare valori, regole e gerarchie, e credo che da qui dovremo andare ulteriormente avanti con una riorganizzazione più generale. Ma la cosa importante, e su questo voglio concludere, è capire fino in fondo le ragioni: non solo cosa è successo nei suoi dettagli, ma perché è successo, chi ha deciso che succedesse proprio questo, per quali esigenze, per quali fini, per quali progetti. possibile, è ancora più importante. Ci vuole chiarezza e trasparenza. Siamo in un momento in cui si fanno mille ipotesi e illazioni: chi parla di gas kazako, chi di servizi segreti. Queste ombre vanno rimosse. A noi non interessa la dietrologia, né le ricostruzioni di fantasia, ma le ombre vanno rimosse: il Parlamento deve sapere su che terreno ci muoviamo e tutto il Paese ha bisogno di essere messo messo trasparentemente a conoscenza di queste cose. Con questi elementi a disposizione credo che anche il dibattito politico potrà essere pienamente libero e all'altezza del compito che è chiamato a svolgere. Mi fermo qui e approfitto di questo intervento per ringraziare, perché in questi giorni è stato svolto da parte del nostro Senato e della nostra Camera un ruolo importante, svolto anche dalla Commissione diritti umani, presieduta dal senatore Manconi, che sin dall'inizio di questa vicenda si è interessato per cercare di

ma anche una caduta sul tema dei diritti non deve mai più accadere. Credo dunque che il contributo offerto dal Senato con i lavori della sua Commissione possa essere apprezzato. Con questi intendimenti e questo modo di vedere le cose ci apprestiamo dunque ai prossimi passaggi di questa vicenda.